negli atti del Senato della Repubblica sarà facile ritrovare più di un sollecito affinché il Governo desse risposta. Essa prendeva spunto da una notizia apparsa il 18 ottobre 2006 sull'agenzia israeliana Debka, che concerneva la presunta vendita di quindici missili terra-aria da parte del Governo italiano al Governo del *premier* libanese Siniora, le cui finalità sarebbero state quelle di impedire a Israele il monitoraggio delle attività terroristiche sul territorio libanese. Dalla lettura dell'interpellanza appare chiaro che la notizia, si potrebbe dire, aveva il valore che Max Weber assegnava all'idealtipo. Era cioè spia di una situazione più complessiva e questa situazione risiedeva nel fatto che della risoluzione 1701 dell'11 agosto 2006, approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la quale è stato previsto il potenziamento del contingente militare UNIFIL,

quella disposizione fosse rispettata anche dagli altri attori della vicenda appariva in qualche modo molto In quei giorni vi erano delle prove che andavano in tal senso. Proprio a quel periodo, infatti, risale un rapporto dell'*intelligence* militare israeliana, che aveva dimostrato, con prove inconfutabili, la cadenza quotidiana delle consegne di armi ai guerriglieri che dal Nord della Siria giungevano a destinazione nel Sud-Ovest del Libano. D'altra parte, sempre in quei giorni, e in particolare l'11 ottobre 2006, un esponente di primo piano di Hezbollah, Nabil Kaouk, aveva dichiarato (la dichiarazione era riportata sul «Corriere della Sera»): «Se l'UNIFIL nei suoi pattugliamenti sul territorio dovesse vedere convogli di armi, potrebbe allora segnalare all'esercito libanese di requisirle. Ma, ne sono certo, nessuno vedrà le nostre armi. Queste, al momento, sono le regole sul campo». E ancora: «Guai se i contingenti internazionali in Libano dovessero venire usati per isolare o condizionare Hezbollah».

Signori del Governo, mi permetterete, visto il tempo trascorso dall'interpellanza, di fare una brevissima cronistoria su questo aspetto, che porti ad aggiornare qualche dato e quindi anche ad aggiornare l'interpellanza. Il 31 gennaio 2007, il *leader* di Hezbollah Nasrallah, intervenendo nella periferia Sud di Beirut, ha dichiarato: «Il futuro d'Israele è la morte».

che Hezbollah mai disarmerà e che anzi continuerà la sua battaglia per destabilizzare il Libano. Poi prende apertamente in giro la comunità internazionale e annunzia che il tribunale dell'ONU che dovrebbe giudicare gli assassini

di comizi o di interventi pubblici nei confronti di quelli che più che seguaci si possono definire fedeli. Tuttavia, dal maggio 2007 queste manifestazioni sono attentamente monitorate dall'ONU. del rapporto ONU del 7 maggio 2007, il segretario generale Ban Ki-Moon, sull'attuazione della risoluzione 1559 che, come voi sapete, signori del Governo, esige il disarmo delle milizie in Libano, sostiene: «Ho ricevuto informazioni da Israele sul traffico d'armi. Tali informazioni sono dettagliate e sostanziali, come descritto nel mio recente rapporto. In più ho ricevuto rapporti da altri Stati membri che dettagliano il trasferimento illegale di armi. Secondo tali rapporti, alcune armi prodotte fuori dalla regione arrivano attraverso Paesi terzi e sono portate clandestinamente in Libano attraverso il confine siro-libanese». Inoltre, nel rapporto, Ban Ki-Moon ricorda una serie puntuale di violazioni, riportate dai notiziari internazionali, denunziate dal Governo libanese, registrate e documentate dal Governo israeliano, dalla stessa UNIFIL e da Paesi terzi e in alcuni casi ammesse esplicitamente da Hezbollah, al punto da annunziare l'invio di un *team* di esperti per verificare la situazione.

l'esplosione che ha colpito, fortunatamente senza gravi conseguenze, il contingente della Tanzania nella zona di responsabilità italiana. In questi giorni e di fronte a questi avvenimenti, il rapporto Libat indica come, come, nonostante l'evidenza lampante di ogni tipo di traffico e di contrabbando, nessuno dei testimoni abbia riportato un singolo incidente di violazione del confine, di qualsiasi tipo.

come il propagarsi delle aree di tensione militare stia mettendo a dura prova l'esercito libanese, sminuendone quindi la capacità operativa nel Sud del Libano. Questo rapporto cita una serie di episodi provati di violazioni delle risoluzioni ONU, sia la 1559 che la 1701, da parte della Siria e soprattutto di Hezbollah e mette in guardia contro nuovi incidenti, indicando la presenza di armi sul territorio sotto il controllo dell'UNIFIL; cita, inoltre, gli attacchi e gli attentati contro obiettivi civili e politici in Libano; cita, infine, il rifiuto di Hezbollah ad adempiere l'obbligo, secondo le risoluzioni 1559 e 1701, di disarmare la propria milizia. Andiamo a tempi ancora più recenti. Vediamo cosa le agenzie, sia nazionali che internazionali, battono il 20 luglio, ovvero qualche giorno fa, sull'incontro che si è verificato a Damasco tra il Presidente dell'Iran Ahmadinejad con i *leader* di Hezbollah Nasrallah e Meshaal. I due *leader*, alla fine dell'incontro, hanno ringraziato il dittatore iraniano e in cambio hanno ricevuto questa dichiarazione: «La e questo ci porta a pensare che il regime sionista si stia indebolendo ogni giorno di più». Queste dichiarazioni, che vengono - ricordo - da un *leader* internazionale che è giunto fino al al punto di negare l'Olocausto e di promuovere nella sua capitale un grande convegno per dimostrare l'inesistenza dell'Olocausto, sono state puntualmente rilanciate, due giorni dopo, dal *leader* libanese Nasrallah, il quale, in un'intervista alla rete televisiva Al Jazeera, ha affermato: «Tel «Tel Aviv o altrove, siamo sicuri di poter raggiungere ogni angolo, ogni luogo della terra della Palestina occupata» - signori del Governo, la terra della Palestina occupata è ovviamente Israele nel linguaggio di Nasrallah di Nasrallah - «Siamo sicuri di poterlo fare». Ecco, questa è la situazione. Avrei altre citazioni di *leader* di Hezbollah, tutte quante mettono in rilievo il fatto che in quest'anno, nel periodo che è intercorso dal momento nel quale la mia interpellanza è stata presentata ad oggi, Hezbollah ha continuato ad armarsi; la sua forza è diventata maggiore di quella di un anno fa e tutto ciò senza che abbia avuto la volontà, o forse la possibilità, di intervenire per evitare che le risoluzioni dell'ONU fossero così palesemente disattese. disattese. Dunque, al di là dell'episodio che è citato nella interpellanza, che - come ho detto all'inizio - può essere considerato quasi un idealtipo

sapere se queste informazioni, che provengono da fonti così diffuse - non solamente fonti giornalistiche ma anche rapporti ufficiali o di organizzazioni internazionali o di istituti specializzati - abbiano un fondamento e quali sono le determinazioni che il Governo sta assumendo affinché

relativa alla possibile vendita da parte del Governo italiano di missili, è completamente falsa; può essere presa come spunto o emblema non so di cosa, ma comunque è una notizia falsa che non ha nessun elemento di fondamento. La missione UNIFIL, come voi sapete, nasce dalla risoluzione 1701 del

forze che in quel momento si contrapponevano, anche attraverso l'uso delle armi, e si potevano considerare forze belligeranti, a partire da Israele, così come dal Libano e anche dal movimento politico di Hezbollah.

600 minori, aveva procurato distruzioni di vario tipo e attacchi con lanci di missili nello stesso territorio a Nord di Israele. di entrata in vigore della tregua e dall'avvio dell'operazione UNIFIL, la tregua tiene, nonostante tutte le difficoltà e le tensioni che rimangono, soprattutto di carattere politico interno condizionato anche da situazioni esterne di particolare gravità. di particolare gravità. Da quel momento non vi è più stato un morto dovuto ad operazioni belliche di questo tipo. Quindi, la risoluzione e la missione UNIFIL sono anche a garanzia di Israele, tanto che, per la prima volta, Israele accetta di assegnare a

su cui è in corso un'indagine, e comunque l'intervento dell'esercito libanese ha consentito che rimanesse un atto completamente isolato.

diventasse operativa attraverso la piena disponibilità data ad intervenire nella missione, ad assumersene eventualmente la responsabilità del comando, cosa che ha consentito di sbloccare anche la partecipazione degli altri Paesi.

che non avveniva - se non ricordo male - da circa 30 anni. Quello, infatti, era uno dei compiti fissati dal Consiglio di Sicurezza.

autorizzava UNIFIL ad adottare «ogni azione necessaria» (incluso quindi anche l'uso della forza) nell'area di dispiegamento esclusivamente in cinque casi chiaramente specificati dalla stessa risoluzione: 1) assicurare che l'area in questione non sia utilizzata per attività ostili di alcun genere; 2) resistere a tentativi volti - attraverso l'uso della forza - ad impedire alla missione di svolgere i propri compiti in base al mandato conferitole; 3) proteggere il personale, le attrezzature, le istallazioni e l'equipaggiamento del personale dell'ONU; 4) assicurare la sicurezza e la libertà di movimento del personale dell'ONU e degli operatori umanitari, fatta salva la responsabilità del Governo del Libano al riguardo; 5) proteggere i civili sottoposti ad imminente minaccia di violenza fisica. Vorrei ricordare che l'UNIFIL agisce in uno Stato sovrano e che, quindi, deve innanzitutto rispettare la sovranità ed il ruolo sia del Governo che dell'esercito regolare di quel Paese.

l'accompagnamento del dispiegamento dell'esercito libanese nel Sud del Paese e lungo la Linea Blu, contestuale al ritiro israeliano; il coordinamento delle attività con i Governi libanese ed israeliano (al riguardo voglio sottolineare che tale coordinamento funziona; a livello militare ci sono riunioni periodiche, non dico presiedute, ma assistite dal nostro comandante della missione sul campo); il sostegno alle attività umanitarie ed al rientro degli sfollati; l'assistenza alle Forze armate libanesi nel prendere misure per lo stabilimento della *buffer

e la Linea Blu; l'assistenza al Governo libanese - su sua richiesta - per controllare i confini al fine di prevenire l'ingresso di armi. UNIFIL, dunque, ha il compito di assistere le Forze armate libanesi nello svolgimento di queste attività a loro a loro stesse assegnate e di rendere l'area compresa tra il fiume Litani e la Linea Blu "libera" da combattenti ed armamenti diversi da quelli delle forze regolari libanesi e della stessa UNIFIL. Da più parti

tra Siria e Libano, e che - così come risulta dai risultati della missione delle Nazioni Unite sull'espletamento della risoluzione

più attuabile e praticabile non è quella di dislocare una forza nazionale lungo il confine tra Siria e Libano, perché probabilmente avremmo bisogno di altre 10.000-15.000 unità non concretamente reperibili e quindi non disponibili, ma quella di individuare individuare un'apposita missione di sostegno, di aiuto, di formazione, di istruzione, insomma di sostegno in senso ampio, all'esercito libanese perché possa migliorare l'efficacia dei controlli su quel confine.

Vorrei intanto precisare preliminarmente che i missili Aster 30, destinati alla difesa aerea a medio raggio, vengono impiegati esclusivamente in combinazione con il sistema di lancio *Soil-Air Moyenne Portée-Terrestre* (SAMP-T). Il citato sistema missilistico, attualmente nella fase di sviluppo, non è stato ancora introdotto nella linea operativa dell'Esercito italiano. L'unica linea di produzione del sistema, realizzato da EUROSAM, un consorzio di società italo-francesi che collaborano con con lo sviluppo dei sistemi della cosiddetta Famiglia Antiaerei Futuri, è ubicata in Francia, mentre in Italia sono costruite soltanto alcune componenti. A tal riguardo, non risulta l'esistenza di trattative tra la citata EUROSAM ed il Governo libanese per la vendita dei predetti sistemi d'arma, che naturalmente non essendo in possesso del nostro Paese non solo non potevano essere dal nostro Paese venduti, ma neanche poteva essere presa in considerazione la possibilità di venderli. Nel contempo, si precisa che non vi sono in atto iniziative per l'invio in Libano di istruttori italiani con il compito di addestrare militari di quel Paese all'impiego dei missili ASTER 30. Per quanto riguarda, più specificatamente, l'attività svolta dal contingente italiano, si fa notare che i nostri militari stanno rispondendo pienamente agli scopi della missione, sviluppando una costante cooperazione con l'esercito regolare del Libano per mettere in atto i meccanismi di coordinamento, affinché UNIFIL possa efficacemente assistere il Governo libanese nell'esercizio della sua sovranità nell'area di operazione. Gli obiettivi sono volti a mantenere un atteggiamento imparziale, così da preservare il consenso delle parti verso la missione e le forze UNIFIL, e prevenire il discredito della missione da parte di fazioni o gruppi ostili; ad aumentare e consolidare la credibilità delle forze UNIFIL e delle forze libanesi schierate nell'area di responsabilità; a promuovere attività ed atteggiamenti miranti a conservare il supporto ed il consenso della popolazione locale.

pensabile che l'intervento della missione da sola possa risolvere la crisi libanese. È chiaro che la missione, garantendo il perdurare di un periodo di tregua, deve servire a dare il tempo alle parti in causa affinché individuino e riescano a realizzare una soluzione politica, perché soltanto attraverso una soluzione politica delle questioni interne al Libano anzitutto e di quelle che riguardano il rapporto tra Libano e Israele si potrà assicurare un periodo periodo di stabilità, di serenità e di pace per quell'area così fortemente martoriata da fenomeni bellici e di violenza. Il Governo Il Governo italiano, lo voglio sottolineare, nei molteplici contatti che intrattiene con i suoi interlocutori libanesi continua ad incoraggiare tutte le forze politiche affinché si impegnino a fermare ogni manifestazione di violenza e a proseguire il dialogo, con l'intento di individuare una soluzione condivisa sui diversi aspetti della crisi, che noi individuiamo nella formazione di un Governo di unità nazionale, nell'elezione di un nuovo Presidente della Repubblica (che, come l'interpellante sa certamente, è prevista a breve), nella nuova legge elettorale e nelle elezioni politiche anticipate. Infine, si fa rilevare che il sequestro avvenuto l'8 febbraio scorso nella periferia di Beirut da parte dell'esercito libanese di un carico di armi la cui proprietà è rivendicata da Hezbollah dimostra la volontà del Governo libanese di rispettare gli impegni ad esso affidati dalla risoluzione n. 1701 con la messa in atto di una decisa azione di contrasto al contrabbando di armamenti e di attrezzature militari. Per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate da Hezbollah, chiaramente sono dichiarazioni che non condividiamo e non sappiamo neanche per quale motivo siano state così ripetutamente citate e riportate da parte dell'interpellante.

mi dichiaro soddisfatto per quello che concerne la risposta sui sistemi d'arma; d'altra parte, era una notizia assunta da una fonte accreditata. Lo scopo delle interpellanze è proprio quello di chiedere al Governo una conferma o una smentita. Mi sembra che la smentita ci sia stata e anche documentata.

In secondo luogo, faccio presente che nessuno ha messo in discussione la risoluzione n. è stata messa in discussione la sua applicazione ed è stato avanzato il sospetto che in realtà

una cosa è la propaganda, altra cosa sono le fonti diplomatiche e cosa ancora diversa è quando tali citazioni vengono riprese puntualmente in rapporti di agenzie internazionali o di istituti

con morti e feriti, e di attentati si susseguono senza fine. D'altra parte, è chiaro, non era possibile ritenere che la situazione si pacificasse in un attimo. Ma il problema,

una situazione che potrebbe ben presto sfociare in qualcosa di peggio di ciò che abbiamo sin qui conosciuto. Sotto questo aspetto, conosciamo

del 22 settembre 2006: «Noi dobbiamo innanzitutto osservare e quindi informare l'esercito libanese. Se noi vediamo qualcosa di pericoloso, informiamo l'esercito libanese il quale deciderà sull'eventuale azione, indipendentemente o concordando con noi le forme di una reazione congiunta». Vorremmo, almeno, che ci si attestasse a ciò ma mi sembra che reazioni congiunte non Capisco che bisogna avere prudenza perché ci sono i nostri uomini e i nostri ragazzi in Libano. Capisco dichiarazioni come quelle rese dal Ministro degli esteri di Hezbollah che dei

l'esigenza di prudenza, ma una cosa è la prudenza, altra cosa è l'efficacia di un'operazione. Se un'operazione dovesse servire solamente come foglia di fico rispetto a ipotesi tendenti al riarmo

la questione su cui alcuni senatori hanno interpellato il Presidente del Consiglio e i Ministri dell'economia e delle infrastrutture è molto delicata e attiene

dell'amministratore delegato di Alitalia, già amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Giancarlo Cimoli e delle indennità di fine rapporto da questi maturate.

l'indennità dei *managers* delle società per azioni pubbliche, si dovesse rispettare un tetto massimo, per le società aventi un impatto sul mercato, di 500.000 euro l'anno, più 250.000 euro l'anno di ulteriore

sia simultaneamente presidente dell'ANAS e presidente della società Stretto di Messina,

sostituire il direttore generale. E chi propone come direttore generale dell'ANAS, di cui è presidente? Naturalmente, propone se stesso che, dunque, diventa anche direttore generale della società di cui è presidente. Gli interpellanti ravvisano in questo una prima violazione, perché non c'è dubbio che sussista un conflitto di interessi quando il controllante presidente la questione è che viene applicato a Ciucci, direttore generale, dal Consiglio di amministrazione la norma della legge finanziaria,

come Presidente; si assume come direttore generale per un tempo di due anni eccedenti la sua carica di presidente. Quindi, quando decadrà da presidente, rimarrà in carica come direttore generale per i due anni successivi.

Ebbene, per quanto questo sia un rapporto di lavoro e non esattamente una funzione manageriale, viene però stabilito per questo rapporto di lavoro il limite dei 500.000 euro più i 250.000. Dunque, l'ingegner Ciucci percepisce queste due somme.

Fatta questa operazione, sembra a noi che nella figura dell'ingegner Ciucci si sommino le seguenti condizioni di natura economica: una indennità in quanto presidente possibilmente anche una indennità in quanto membro del Consiglio di amministrazione. Per quello che se ne sa dalle passate gestioni, nel Consiglio di amministrazione dell'ANAS si percepiva un'indennità come consigliere e poi un'indennità speciale come presidente e quindi potrebbero esserci queste due indennità. Poi ci sono i 500.000 euro

essi vengono poi annualmente fissati. Contemporaneamente a questo, l'ingegner Ciucci sembra assommare su di sé anche l'indennità di presidente della società Ponte sullo Stretto.

il presidente, il vice presidente e l'amministratore delegato della società Stretto Zamberletti, Bucci e Ciucci. Bucci, tra l'altro, è vice direttore generale dell'ANAS, perché Ciucci, andando in ANAS, ha preso Bucci, vice presidente della società Stretto di Messina, e lo ha nominato suo vice direttore.

Ammettendo, quindi, che il presidente, l'amministratore delegato e il vice presidente percepiscano più o meno la stessa cifra, è facile immaginare che circa 350.000-400.000 euro siano imputabili alla figura dell'amministratore delegato, che delle tre è sicuramente quella meglio remunerata.

Allora, noi chiediamo se questo sia vero e cosa risulti dell'insieme dei dati e, nel caso ciò sia vero, che cosa si voglia fare per venire a capo di questa situazione. Chiediamo altresì di sapere cosa si voglia fare nei confronti del rappresentante della Corte dei conti presso l'ANAS e del presidente del Collegio sindacale dell'ANAS, che hanno tacitamente approvato questa situazione che - a nostro giudizio - rasenta

con l'interpellanza in oggetto il senatore Paolo Brutti e altri pongono quesiti in ordine agli organi amministrativo e di controllo dell'ANAS. sentita anche la citata società, si fa presente che il 20 luglio 2006 l'assemblea dell'ANAS ha nominato il dottor Pietro Ciucci presidente della società per un triennio, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008. Il 27 luglio 2006 il consiglio di amministrazione dell'ANAS, ai sensi dell'articolo 182 dello statuto sociale, attribuiva al dottor Ciucci le deleghe in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato al consiglio dallo statuto stesso. Il 21 settembre 2006 il consiglio di amministrazione deliberava di instaurare un rapporto di lavoro dipendente con il dottor Ciucci e, tenuto conto, tra l'altro, delle raccomandazioni espresse dall'azionista nell'assemblea del 20 luglio, deliberava, con l'astensione del dottor Ciucci, di attribuire allo stesso, con effetto immediato, la carica di direttore generale, ai sensi dell'articolo 24 dello statuto sociale. La nomina a direttore generale non richiedeva l'attribuzione di ulteriori deleghe al dottor Ciucci, considerate quelle già attribuitegli ai sensi dello statuto sociale nella qualità di presidente. Tale nomina è del tutto legittima in base allo statuto e a quanto previsto dalla normativa in vigore; essa è finalizzata a obiettivi di semplificazione organizzativa e di efficacia dell'azione aziendale. La retribuzione annua lorda del dottor Ciucci, nei limiti dell'articolo 1, comma 466, della legge finanziaria 2007, ammonta a euro 500.000, oltre ad una quota variabile nella misura del 50 per cento della retribuzione stessa, che maturerà al raggiungimento di obiettivi annuali, possibilmente correlati al piano industriale. È stato inoltre previsto il mantenimento delle coperture preesistenti in tema di previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e polizze assicurative. Il trattamento riconosciuto dal consiglio d'amministrazione al dottor Ciucci è unico per l'incarico di presidente, direttore generale e consigliere d'amministrazione e ricomprende anche i compensi relativi ad eventuali incarichi conferiti dall'ANAS in società controllate e partecipate. Non c'è quindi una remunerazione aggiuntiva. Sulla questione si fa preliminarmente presente che il contratto di lavoro dirigenziale del dottor Ciucci non è quinquennale ma a tempo indeterminato, in quanto connesso al rapporto di amministrazione, il cui venir meno determina anche la risoluzione del contratto di lavoro stesso. La corresponsione dell'importo *una tantum* di 312.500 euro, relativo al periodo 27 luglio-28 dicembre 2006, a valere sul rapporto di amministrazione, è stata deliberata nel pieno rispetto della procedura prevista dall'articolo 2389, comma 3, del codice civile, compreso il prescritto parere del collegio sindacale. Questo importo riguarda un periodo di cinque mesi non coperto dal contratto di lavoro dirigenziale, nel corso del quale il dottor Ciucci ha esercitato pienamente tutte le sue funzioni senza alcuna remunerazione. Nella delibera di nomina a direttore generale della società non trova applicazione l'articolo 2389, comma 3, del codice civile, in quanto, come la giurisprudenza ha chiarito (tra le altre, la sentenza della Cassazione, sezione lavoro, n. 8279 del 10 novembre 1987), qualora nella stessa persona si cumulino le funzioni di amministratore e di direttore generale, si instaurano due distinti rapporti, rispettivamente di amministrazione e di lavoro subordinato. Mentre il rapporto di lavoro subordinato è regolato dal contratto collettivo di lavoro della categoria cui appartiene il lavoratore, solo per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche trova applicazione l'articolo 2389, comma 3, del codice civile e solo tale situazione è disciplinata dal comma 466 della finanziaria 2007, procedura seguita per remunerare il periodo 27 luglio-28 dicembre 2006, in cui il Presidente ha operato come amministratore investito di cariche operative in virtù delle deleghe conferitegli dal consiglio. contratto di lavoro dipendente stipulato il 28 dicembre 2006, ancorché non soggetto alle disposizioni di cui al comma 466 della finanziaria 2007, che sono, tra l'altro, entrate in vigore il primo gennaio 2007, si è comunque uniformato per la parte economica, d'intesa con l'azionista, ai criteri previsti dal citato comma, mentre per la parte normativa fa riferimento al contratto nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'ANAS. Relativamente all'incarico di amministratore delegato della società Stretto di Messina, è stato previsto fin dalla stipula del contratto con ANAS che il compenso dovuto *ex* articolo 2389, commi 1 e 3, del codice civile, peraltro dimezzato a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia riversato, a seguito di rinuncia da parte del dottor Ciucci, da Stretto di Messina ad ANAS, in quanto l'incarico, essendo ricoperto dal maggio 2002, era precedente a quello di presidente e direttore di ANAS. L'impegno del dottor Ciucci a tale rinuncia risulta dal libro verbali del consiglio di amministrazione di Stretto di Messina Spa. In proposito, si fa presente che anche in passato i compensi di cui trattasi venivano versati direttamente da Stretto di Messina a Fintecna, precedente datore di lavoro del dottor Ciucci. Si precisa, inoltre, che a seguito del trasferimento ad ANAS, così come stabilito dal comma 92 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, del pacchetto azionario di controllo della società Stretto di Messina, nell'autunno 2007 si darà luogo alla nomina di un nuovo amministratore delegato. Si soggiunge che gli incarichi di collaudatore di alcune opere parziali nell'ambito del progetto MOSE, nonché di consigliere della Banca popolare di Roma sono a loro volta antecedenti alla nomina del dottor Ciucci a presidente della società ANAS, prevedono compensi di ridotta entità e non configurano conflitti d'interesse con ANAS. Per quanto riguarda il riferimento al comma 593 della legge finanziaria 2007, si precisa che nella fattispecie non trova applicazione, in quanto la norma citata si riferisce ai dirigenti della pubblica amministrazione e non a quelli di società per azioni, ancorché con capitale di maggioranza pubblica. Nei termini suesposti è stata svolta l'attività del collegio sindacale *pro tempore*, che si ritiene abbia operato correttamente, nel rispetto delle disposizioni civilistiche e statutarie. Si precisa che, ai sensi del comma 3, dell'articolo 2389 del codice civile, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, non essendo quindi prevista alcuna competenza da parte degli azionisti. Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze ha esplicitatamente affermato di non esercitare attività di direzione e coordinamento nei confronti delle proprie partecipate, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile. Con riferimento alla posizione del dottor Parlato citata dagli interroganti, si precisa che egli fino al 19 luglio 2007 ha rivestito la qualifica di dirigente dell'ufficio che, nell'ambito della Direzione finanza e privatizzazioni del Dipartimento del tesoro, ha avuto la responsabilità dei processi di privatizzazione delle partecipazioni dello Stato e, inoltre, ha supportato la direzione nel monitoraggio, controllo e esercizio dei diritti dell'azionista delle società di competenza (società quotate e Fintecna). Solo dal 20 luglio scorso egli ha ricevuto l'incarico di responsabile della Direzione generale finanza e privatizzazioni del Dipartimento del tesoro con conseguente ampliamento delle proprie competenze alle società controllate dallo Stato. Nell'ambito delle funzioni precedentemente svolte, egli non ha avuto alcuna competenza su ANAS, società rientrante nelle attribuzioni di un altro ufficio della Direzione. Con riferimento alla società Stretto di Messina, quest'ultima è una partecipata di secondo livello dello Stato, essendo controllata da Fintecna, ANAS e FS, oltre che dalle Regioni Calabria e Sicilia. Proprio per il controllo indiretto della società, il Ministero dell'economia e delle finanze negli ultimi anni ha avuto un coinvolgimento limitato ad iniziative connesse

disposto dall'articolo 23 commi 91, 92 e 93 della legge n. 286 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 262 del 2006, quale atto propedeutico al versamento da parte di Fintecna allo Stato delle risorse a suo tempo destinate al progetto Ponte sullo Stretto sullo Stretto (1,5 miliardi circa, oggetto di delibera assembleare nel 2004 e non versati alla Società Stretto di Messina).

dalla situazione descritta dagli interpellanti deriva uno stato di forte preoccupazione, mentre apprendo che il Governo la trova invece una situazione del tutto legittima. Di questo prendo atto, anche se seguito a non essere d'accordo, né soddisfatto.

euro, tenuto conto che l'ANAS ha chiuso il bilancio dell'anno scorso in passivo, chiude il bilancio di quest'anno in passivo, si prevede che chiuderà il bilancio dell'anno prossimo in passivo e che solo dal 2009

il conflitto d'interessi, invece, mi dichiaro insoddisfatto dell'osservazione che viene fatta, perché credo che la funzione di direttore sia una cosa (e infatti è lavoro dipendente) e la funzione di presidente o di amministratore delegato sia un'altra cosa, e ritengo che tra le due funzioni vi sia un rapporto di vigilante-vigilato

infrastrutture*. I PRUSST, ovvero i Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, sono stati promossi con il decreto ministeriale del 8 ottobre 1998 recante «Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio"». Gli obiettivi del programma, così come riportati dall'articolo 2 del decreto, sono i seguenti: la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, avuto riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico e garantendo l'aumento di benessere della collettività; la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all'ampliamento e alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali e artigianali, alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado. Per quanto attiene quindi al sistema di valutazione dei programmi e progetti presentati, si precisa che l'amministrazione, attraverso la pubblicazione del bando allegato al citato decreto 8 ottobre 1998, ha fissato le norme per partecipare ai programmi, i criteri di valutazione e il finanziamento. L'articolo 5 del bando prevedeva che le proposte ai soggetti promotori venissero formulate dai seguenti soggetti proponenti: enti pubblici territoriali (Regione, Province, comunità montane); altre amministrazioni pubbliche (le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo); le istituzioni universitarie; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; le società e le imprese a partecipazione pubblica; gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati; denominati; soggetti privati (associazioni di categoria, imprenditori, società finanziarie, istituti bancari proprietari degli immobili, soggetti concessionari, proprietari o gestori di rete). I soggetti proponenti hanno inviato delle proposte ai Comuni i quali hanno promosso i programmi in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, ove esistenti, e hanno assicurato l'integrazione e la concertazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio. Previa intesa con i Comuni interessati, i programmi sono stati promossi anche da Province e Regioni. Ai fini dell'individuazione degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 3, comma 1 del citato decreto (assi prioritari d'intervento), i soggetti promotori hanno favorito la più ampia partecipazione all'attuazione dei programmi da parte di soggetti pubblici e privati; è inoltre competenza dei soggetti promotori la verifica della compatibilità e la coerenza dei programmi con le indicazioni dei documenti di pianificazione urbanistica e territoriale. A tal fine, il bando allegato al decreto ministeriale del 1998 (articolo 8) disponeva che i soggetti promotori dei programmi trasmettessero la documentazione relativa ai progetti alla Direzione generale per il coordinamento territoriale (DICOTER) del Ministero dei lavori pubblici e alla Regione competente per territorio entro sei mesi dalia data di pubblicazione del bando avvenuta il 27 maggio 1999. Tali termini sono stati poi prorogati al 27 agosto 1999, stabilendo inoltre che la sottoscrizione degli accordi-quadro avvenisse entro il mese di dicembre 2000 (decreto ministeriale del La valutazione dei programmi da ammettere a finanziamento è stata effettuata da un «Comitato di valutazione e selezione», istituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, composto da: un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzione di Presidente; quattro rappresentanti designati da amministrazioni centrali dello Stato; quattro rappresentanti designati dalla Conferenza unificata; un rappresentante designato da ciascuna Regione. I programmi, conformi agli obiettivi e ai requisiti generali indicati nel bando, sono stati quindi valutati sulla base dei seguenti criteri: capacità di attrarre investimenti produttivi e di sviluppare iniziative economiche e imprenditoriali in grado di garantire una ricaduta socio-economica positiva stabile e duratura,

metodologie progettuali e di intervento qualitative basate su logiche di risultato e, dall'altro lato, tecniche finanziarie innovative anche nell'utilizzo di risorse pubbliche; presenza di interventi pubblici, realizzati con risorse esclusivamente private, che prevedono corrispettivi di gestione; presenza, nell'ambito territoriale considerato, di indicazioni circa l'avvio di rilevanti fenomeni di sviluppo economico e di trasformazione territoriale; rapidità di implementazione delle azioni e delle iniziative previste nei programmi in relazione alla copertura finanziaria

gli elementi di criticità legati al rapporto infrastruttura-sistema urbano in termini territoriali e ambientali; congruenza dei programmi con piani/politiche di settore nazionali e regionali. La valutazione dei programmi è stata finalizzata all'attribuzione di un punteggio complessivo di 100 punti, così ripartito. 80 punti assegnati in base ai seguenti indicatori: capacità dei programmi di garantire l'integrazione tra politiche settoriali (40 punti), misurata sulla base degli importi finanziari finalizzati alle politiche di recupero del *deficit* infrastrutturale; alle politiche di recupero, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio ambientale; alle politiche che perseguono fini sociali, per insediare attività produttive in grado di garantire effetti occupazionali stabili e alle politiche di partenariato di sussidiarietà e di concertazione locale; capacità concertazione locale; capacità dei programmi di implementare le azioni e le iniziative previste in relazione alla copertura finanziaria, 20 punti, misurata sulla base dei finanziamenti già disponibili sul totale della provvista necessaria, percentuale dell'investimento da parte dei soggetti privati che partecipano all'attuazione dei programmi superiore ad un terzo dell'investimento complessivo e degli interventi pubblici realizzati con risorse parzialmente o integralmente private; private; capacità dei programmi di rispondere alle esigenze espresse (qualità della progettazione), cui venivano attribuiti 20 punti, misurata sulla base della presenza significativa di obiettivi programmatici per quanto attiene alla qualità ecologica, alla qualità urbanistica e alla qualità morfologica o dei tessuti urbani; la previsione di interventi chiaramente orientati ai seguenti settori: ambiente, paesaggio, accessibilità e sicurezza del territorio, equipaggiamento e dotazione di servizi, complessità morfologica e dei tessuti urbani; presenze significative di approfondimenti progettuali nei seguenti settori: valorizzazione ed emergenze naturali, eliminazione dei fattori ambientali, recupero e valorizzazione delle emergenze antropiche, uso della vegetazione a scopo paesaggistico, integrazione con la rete veicolare esterna, localizzazione strategica dei parcheggi, continuità e indipendenza della rete pedonale e ciclabile, sicurezza e protezione degli spazi aperti, attrezzature a compenso del contesto, flessibilità e polifunzionalità dei servizi, recupero fondiario ed edilizio, assortimento tipologico, conservazione e valorizzazione delle tipologie speciali. Ulteriori 20 punti sono stati assegnati sulla base degli indicatori stabiliti da ciascuna Regione per l'ammissione a finanziamento dei programmi localizzati nei rispettivi ambiti territoriali. L'articolo 8, comma 8, del bando allegato al decreto ministeriale dell'8 ottobre 1998 ha inoltre stabilito che, per garantire una efficace azione di coordinamento tra i soggetti interessati alla composizione ed alla realizzazione dei programmi, nonché per pervenire alla sottoscrizione del protocollo d'intesa e alla conclusione dell'accordo-quadro, presso la direzione generale del coordinamento territoriale venisse istituito un tavolo permanente di concertazione, presieduto dal direttore generale o da un suo delegato ed assistito da una segreteria tecnica per la gestione del medesimo. Il protocollo d'intesa rappresenta l'atto con il quale tutte le parti coinvolte nei procedimento si sono impegnate all'attuazione del programma e degli adempimenti che il decreto ministeriale istitutivo richiedeva per la sottoscrizione dell'accordo-quadro. Il passaggio tra il protocollo d'intesa e l'accordo-quadro presupponeva che al promotore ed ai partecipanti al programma fossero ben chiari gli effetti giuridici degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo d'intesa. Alla base del protocollo d'intesa del PRUSST vi era senza dubbio l'accordo tra amministrazioni pubbliche, tra loro autonome, e i privati cointeressati ad un più celere e definito svolgimento dei loro compiti istituzionali. L'accordo quadro del PRUSST è passato attraverso lo strumento del tavolo-di concertazione. Ad ogni tavolo permanente di concertazione ha partecipato un rappresentante del soggetto promotore, un rappresentante della Regione ed un soggetto in rappresentanza dei privati proponenti; il presidente aveva comunque la facoltà di invitare ogni altro soggetto pubblico o privato coinvolto nel PRUSST. Gli impegni che i soggetti sottoscrittori dell'accordo hanno riassunto sono: l'approvazione del programma degli interventi inseriti nel PRUSST; l'individuazione del livello di progettazione degli interventi pubblici; l'approvazione del quadro finanziario e del cronoprogramma relativo all'attuazione degli interventi; l'impegno a formalizzare le predette approvazioni nei modi di legge, con atti della propria amministrazione. Per quanto attiene allo stato di attuazione dei PRUSST, si allega un prospetto recante la situazione dei finanziamenti, suddiviso Regione per Regione, aggiornato al 31 dicembre 2006. Relativamente, quindi, alla richiesta di una eventuale verifica dei progetti realizzati e del preesistente stato dei luoghi, si fa presente che l'articolo 8 dell'accordo quadro sottoscritto per ogni programma, prevedeva l'istituzione di un collegio di vigilanza, composto dal provveditore alle opere pubbliche, dal legale rappresentante del soggetto promotore, dal legale rappresentante della Regione e da due rappresentanti, di cui uno designato dall'assemblea dei soggetti pubblici e l'altro dall'assemblea dei soggetti privati partecipanti al programma. Tale collegio è istituto allo scopo di vigilare sulla tempestiva e corretta attuazione dell'accordo; individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione; provvedere, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito all'attuazione dell'accordo; approvare le eventuali modifiche al programma nonché il rendiconto finale dell'iniziativa. In tutti quei casi in cui venissero rilevate dagli organi preposti alla vigilanza atti impropri nell'individuazione degli interventi e nella conseguente attuazione dei programmi, il Ministero delle infrastrutture garantisce il proprio supporto nei limiti disposti dall'accordo quadro anche attraverso il proprio rappresentane nel Collegio di vigilanza. Per quanto attiene allo stato di attuazione dei PRUSST, si allega un prospetto recante la situazione dei finanziamenti, suddiviso Regione per Regione, aggiornato, come ho detto poc'anzi, al 31 dicembre 2006 facendo presente che i soggetti promotori dovranno fornire gli aggiornamenti relativi ai progetti di propria competenza entro il prossimo mese di agosto per il previsto monitoraggio semestrale. Non risulta, infine, al Ministero che vi siano state procedure di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia.

questo strumento è un'arma che produce effetti negativi sul territorio devastanti per come viene usato. Lei deve sapere, forse meglio di me, che questo strumento, cioè il PRUSST, è anche variante di piano

deroga, con il PRUSST che ha funzionato anche come variante di piano per costruire supermercati di svariate migliaia di metri quadrati di superficie che poi

di circa 450 milioni di euro dati alle varie Regioni che sono finiti, probabilmente, solo nelle mani di professionisti. Io le chiedo - questa era la

soldati che partono per la guerra e non ritornano più. Il Governo ha il dovere di seguirli e di farci capire cosa è accaduto sul territorio e quali effetti

programmazione, come si dovrebbe fare, ma, di volta in volta, a seconda dell'amico imprenditore, intervengono sul territorio,

le competenze del Ministero delle infrastrutture in materia di finanziamenti per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati discendono dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, che prevede la rotazione di contributi agli aventi diritto attraverso la Regione. Sebbene le Regioni continuino ad avanzare richieste di finanziamento per un importo complessivo superiore ai 100 milioni di euro, la legge n. 13 del 1989 è stata finanziata solo fino all'anno 2001. IlMinistero delle infrastrutture, nella Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, negli anni successivi al 2001 ha proposto il rifinanziamento della legge in questione per fare fronte agli impegni derivanti dalla stessa nei confronti della Regione. Tali proposte di rifinanziamento, che non hanno tuttavia trovato accoglimento nelle relative leggi finanziarie degli anni scorsi, verranno reiterate per il prossimo esercizio finanziario, garantendo l'impegno del Ministero in tal senso.

la metto nelle sue mani, signor Vice ministro, alla sua coscienza e a quella del Governo. È dal 2004 che non si eroga più una lira ai soggetti disabili.

alcuna risorsa per garantire la vivibilità, la dignità di vita a persone disabili che non sanno come muoversi, per fare un ascensore che le possa portare al piano, per rivedere i bagni delle abitazioni affinché siano consoni alle loro esigenze.

in direzione di queste categorie, che hanno bisogno e vi chiedono aiuto. Ci sono migliaia di domande da parte di queste persone. Un Governo che non si preoccupa di queste cose, a mio giudizio un Governo non è, e non può essere chiamato tale.

Presidente, con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, il senatore interrogante chiede di sapere quali iniziative questo Ministero intenda assumere a sostegno della creazione del Politecnico veneto, proposta dal rettore dell'Università degli studi di Padova, della quale istituzione peraltro il Ministero non conosce alcun dettaglio tecnico. Devo sottolineare in merito che l'istituzione di nuovi atenei, statali o non statali legalmente riconosciuti, è definita nell'ambito delle procedure relative alla programmazione triennale del sistema universitario.

La nuova normativa innova sensibilmente quella previgente, sia nel metodo che nelle procedure da attuare per la definizione delle linee generali di indirizzo per il sistema universitario per ciascun triennio.

attualmente alla Corte dei conti per la registrazione, con il quale sono state definite le linee generali di indirizzo per la programmazione delle università per il triennio 2007-2009. Nel predetto provvedimento si fa presente che, considerata l'entità delle risorse disponibili per il sistema universitario e l'opportunità che le stesse siano interamente impegnate per le università esistenti, nel corso degli anni 2007, 2008, 2009 non si darà corso alla istituzione di nuove università statali. Non si esclude peraltro che, in provvedimenti di legge attualmente allo studio sulle forme e procedure di governo del sistema universitario nazionale e delle singole università, non possano essere individuate nuove procedere per l'istituzione di nuove università, anche tramite la suddivisione di esistenti, che dovrebbero comunque prevedere: la valutazione stringente, da parte dell'istituenda Agenzia nazionale di valutazione, della sostenibilità culturale, didattica, scientifica, tecnologica, infrastrutturale e, naturalmente, finanziaria dell'iniziativa; inoltre, la compartecipazione decisionale ed eventualmente finanziaria degli enti territoriali e dei sistemi sociali interessati; e, infine, l'accordo dei corrispondenti sistemi universitari regionali. In questo quadro, l'ampliamento del sistema nazionale dei politecnici, attualmente comprendente solo i politecnici di Bari, Milano e Torino, potrà essere riconsiderato con l'obbiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo tecnologico del Paese.

di costituire un sistema a rete tra gli istituti e i poli di ricerca già esistenti all'interno delle Università di Padova, Verona, Venezia "Ca' Foscari" e l'Istituto di architettura e urbanistica di Venezia. il riferimento alla normativa che esclude l'istituzione di nuove università statali nel territorio nazionale non possa essere preso in considerazione con riguardo alla fattispecie in esame. Resto stupefatto anche del fatto che il Ministero non sia a conoscenza dei dettagli di questo progetto, perché esso è stato presentato con grande enfasi, attraverso un un riscontro mediatico molto efficace, ancora nei mesi di gennaio e febbraio scorso, e quindi non mi capacito di come in realtà non sia ancora arrivato nella stanza dei bottoni al Ministero. La sua risposta di oggi, onorevole Sottosegretario, è peraltro anche l'occasione per il sottoscritto di fare un po' il punto della situazione sul tema e mi consente di esprimere alcune valutazioni sul progetto del professor Milanesi che riguarda il Veneto. Innanzi tutto, ritengo molto positivo che i quattro atenei veneti tendano a superare quella logica campanilistica che troppo spesso anche in Veneto ha comportato dispersione di risorse ed inefficienze in tanti settori e che si tenda a creare un polo di eccellenza in grado di competere con i più prestigiosi istituti internazionali di ricerca. Ma per cogliere questo obiettivo si deve evitare che il progetto nasca già vecchio. C'è innanzi tutto un punto della proposta del professor Milanesi che, a giudizio di chi parla, merita di essere discusso con attenzione: mi riferisco al senso che vogliamo dare all'espressione "politecnico". I nomi contano, e in questo caso portano con sé una storia importante. In Italia e in Francia il nome "politecnico" qualifica istituzioni prestigiose che dall'Ottocento in poi hanno contribuito allo sviluppo della scienza e della tecnologia in stretta collaborazione con il mondo delle grandi imprese industriali. I politecnici sono le istituzioni che hanno formato i tecnici su cui l'industria moderna ha potuto contare per sviluppare i cicli continui e le catene di montaggio. Ma mi domando: serve oggi al Veneto una scuola politecnica di tipo tradizionale? Mi sentirei di rispondere negativamente, e non solo perché il nostro è un capitalismo di piccole e medie imprese: la formula del politecnico del futuro dev'essere necessariamente diversa da quella del passato, perché nel frattempo il mondo ha cambiato direzione. È cambiata la percezione che oggi abbiamo della tecnologia e anche il valore che ad essa attribuiamo. Il successo dei prodotti dell'industria è legato certamente all'innovazione tecnologica, ma è legato anche a fattori come l'estetica, il *marketing* e il *design.* Oggi l'innovazione nasce soprattutto dalla riscoperta della centralità della persona: dunque, non solo funzioni, ma anche valori estetici e rispondenza a richieste sociali. La tecnologia da sola non paga, se non è accompagnata da un progetto culturale: esempi come le scarpe Geox, i jeans Diesel, le tute motociclistiche Dainese, la nuova "500" della FIAT ce lo testimoniano. Le aziende citate sono oggi il punto di riferimento di un nuovo modo di pensare il *made in Italy* su scala internazionale. Date tali premesse, l'idea che mi sento di proporre oggi è quella di una scuola politecnica veneta di nuova generazione, che punti ad un originale *mix* tra l'innovazione tecnologica ed una riflessione culturale capace di coniugare ricerca scientifica d'avanguardia ed elementi di cultura umanistica, con un approccio autenticamente multidisciplinare. Insomma, un politecnico di nuova generazione, con una classe docente giovane, motivata e capace davvero di competere sul mercato. Secondo punto: oggi le piccole e medie imprese sono i veri motori dell'innovazione. Le grandi imprese sono molto più conservatrici e spesso preferiscono fare *shopping* di tecnologie elaborate da altri. Innovare significa quindi progettare nuovi mondi e nuovi prodotti, non ottimizzare soluzioni tecnologiche preesistenti. Allora, un collegamento tra il nuovo istituto e il tessuto industriale veneto, che è formato prevalentemente da piccole e medie imprese, è davvero opportuno e necessario. Sotto tale aspetto, mi pare un po' miope la posizione assunta dal presidente degli industriali veneti Riello, che sulla stampa, a fronte del progetto, si è limitato a domandarsi chi sosterrà i costi dell'operazione, quasi che il finanziamento del sistema formativo locale non fosse tema che necessariamente riguarda anche il mondo delle imprese. Se ai positivi esempi di stampo anglosassone vogliamo ispirarci, il rapporto tra scuole di eccellenza e imprese locali è proprio uno dei cardini del sistema di formazione dei *manager* e degli scienziati del domani. Concludo con l'augurio che il dibattito che oggi abbiamo sinteticamente svolto possa essere di stimolo perché questo grande progetto culturale possa trovare nuove concrete possibilità di realizzazione. PRESIDENTE.

Detta interrogazione è stata presentata a seguito della sentenza n. 4266 del 10 maggio 2007 del TAR del Lazio, che ha riconosciuto che i dipendenti interessati dall'istituto della dirigenza sarebbero titolari di un interesse legittimo all'attivazione del dispositivo di legge che prevede l'istituzione dell'area separata della vice dirigenza a partire dalla tornata contrattuale 2006-2007, configurandosi come atto dovuto da parte delle amministrazioni riconducibile a precisi obblighi di legge.